Vi prego di prendere posto,

***Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri,

allo svolgimento di una seduta, peraltro in diretta TV, sulla quale è inutile soffermarsi come importanza. Sono sicuro che in questa occasione non vi sarà, da parte di alcun senatore, motivo di disturbo al civile e ordinato confronto che ci si aspetta in casi come quello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 grazie. vorrei dire amato, senza distinzioni di colore politico, come dimostra la sua carriera con Governi di centrodestra o di centrosinistra. Avrete capito che sto parlando del generale di corpo d'armata Claudio Graziano, che è stato trovato morto nella sua casa. Nato nel 1953, aveva iniziato la sua carriera nell'Accademia militare nel 1972. Era ufficiale degli alpini già nel 1974 ed ha comandato numerose missioni all'estero, in particolare come *force commander* e come rappresentante delle Nazioni Unite in Libano, dal 2007 al 2009. In quell'occasione, da Ministro della difesa ebbi l'onore e il piacere di conoscerlo e, anche dopo essermi consultato con l'allora Presidente della Repubblica, che mi diede conforto nella scelta che stavo per fare, lo nominai prima come mio capo di gabinetto e subito dopo Capo di stato maggiore dell'Esercito;

presidente del Comitato militare dell'Unione europea fino al 2022 ed era adesso presidente del consiglio di amministrazione di Fincantieri. Claudio Graziano era un uomo si dice spesso delle persone che sono venute a mancare, ma in questo caso la mia è una testimonianza veramente diretta e personale - eccezionale,

nel profondo turbamento che aveva ingenerato in lui la scomparsa di Marisa, la sua amata moglie, e che ci aveva visto consapevoli della sua difficoltà, avremmo potuto fare qualcosa di più per stargli vicino. È un dubbio che molti si porteranno, ma in casi come questo l'incommensurabile profondità del dolore dell'animo umano rende difficile immaginare come si potesse intervenire. Oggi noi possiamo solo rimpiangerlo, ricordarlo e, pensando ai suoi pochi familiari - a Roma era un uomo solo, e questo ha pesato molto - e ricordandolo a chi gli ha voluto bene, dedichiamo a lui qualche attimo di raccoglimento.

Signor Presidente, signora Ministra, dichiaro il mio voto contrario a questo disegno di legge costituzionale

Sono motivi che prescindono totalmente dalla questione dei senatori a vita e anche dalla questione, che è stata peraltro autorevolmente sollevata da più parti, di un possibile eccesso di concentrazione di potere. Il mio voto contrario è essenzialmente basato su due motivazioni. La prima: sono contrario perché questa riforma non conseguirà i risultati che lodevolmente si propone attività di governo più efficace e più stabile - ma temo risultati opposti. La seconda: non determinerà il desiderato riavvicinamento tra i cittadini e la politica, ma a mio parere contribuirà a un ulteriore allontanamento. In termini telegrafici, sul primo punto mi sono soffermato il 21 maggio. La riforma sembra non guardare al mondo che ci circonda, dove vicino a noi, in Francia, e al di là dell'Atlantico, ci sono le due Repubbliche nelle nelle quali il capo del potere esecutivo è eletto direttamente dal popolo e - certamente non solo per questa ragione -sono le due repubbliche strutturalmente più in crisi. Inoltre, la riforma non consentirebbe più quei gradi di flessibilità nel sistema che a volte si sono dimostrati utili in situazioni di emergenza in Italia e altrove. Per quanto riguarda la seconda ragione, non credo che avvicinerà i cittadini alla politica - e lo dico con molto rammarico - perché non è una riforma fatta nell'interesse dei cittadini: è una riforma fatta nell'interesse della categoria dei politici, per la quale ho molto rispetto. rispetto. I cittadini, se il Governo sarà meno stabile e meno efficace, contrariamente alla volontà della riforma, saranno penalizzati, mentre vedranno facilmente che si vuole anche in questa corporazione, dopo che in tante altre, dare una tessera di ingresso che è l'elezione a membro del Parlamento, che non è necessariamente un titolo di capacità di governo.

siamo fermamente contrari a questa riforma per tre ordini di ragioni: nel merito, nel metodo e per le conseguenze politiche che avrà. Nel merito, di cui credo si sia parlato molto, in linea di principio mi sembra che questa riforma dica che, se un Governo va male e perde dei cittadini, il *Premier* è comunque blindato, nonostante tutto, qualunque cosa accada al Paese. All'inefficacia della politica si risponde, con una politica più efficace, ma blindando la politica anche quando è inefficace. Potrei dire che basta guardarsi intorno: o siamo i più intelligenti di tutti - cosa su cui, dal punto di vista istituzionale, ho un dubbio - o forse ci dovrebbe sorgere perplessità per il fatto che intorno a noi nessuno lo usa. Si potrebbe dire che la legge elettorale che verrà associata avrà e porterà squilibri che probabilmente la renderanno anche non costituzionale, o comunque che questo è un punto delicato. Si può dire tutto questo, ma nel merito anche voi sapete che questa riforma non funziona. Sapete anche voi - o almeno una grande parte delle persone che sono in quest'Aula a mio avviso, il punto non è questo; non è questo che interessa ed è forse il fatto più negativo. Quello che interessa è il metodo: arrivare a un confronto frontale, sempre e comunque. Ne conoscete rischi e sapete che questo - lo abbiamo già vissuto - può portare a dolorose sconfitte. Ma il punto non è questo, a mio avviso. Il punto è spostare l'attenzione. l'attenzione. Se 120.000 giovani se ne vanno dall'Italia; se 4 milioni di cittadini sono sotto la soglia di povertà; se si ha una situazione per la quale la scuola oggi prepara molto meno che in tutti gli altri Paesi europei,

il bene e il male. Possiamo già dire cosa succederà i prossimi mesi, perché l'abbiamo già visto: diremo che, da un lato, c'è la pulsione verso tragici passati e, dall'altro lato, ci sono i traditori della volontà popolare e andremo avanti così, finché a votare rimarrà

che il prossimo anno noi segheremo un altro pezzo del ramo su cui siamo seduti tutti insieme, cioè le istituzioni repubblicane. Lo faremo con un conflitto continuo, costante, su tutto, che non produrrà niente e al termine di tutto questo saremo tutti più deboli. Io non so se vincerete voi o se vinceremo noi, non ne ho idea; è tutto molto imprevedibile ed effimero. So, però, che più cittadini si allontaneranno dalla politica e se ne allontaneranno talmente tanti che, alla fine, il pericolo democratico sarà non la riforma in sé, ma ciò che essa provoca, ciò che il modo di portarla avanti provoca, ciò che questo modo di discutere della Costituzione provoca. Quello che provoca è la sensazione nel Paese che in queste Aule discutiamo di cose lunari, perché sappiamo perfettamente che i poteri del Presidente del Consiglio sono enormi e le cose che non funzionano sono la pubblica amministrazione, il federalismo

come quelle che sono successe e ne succederanno altre, che i cittadini giudicheranno riprovevoli e non ce ne importerà niente, perché il punto non è riportare i cittadini al voto. Il punto è che a votare rimangano solo le curve perché, se a votare rimangono solo le curve, quello che fai o non fai, quello che produci o non produci diventa irrilevante, perché l'unica cosa che diventa rilevante è il tifo. Il problema è che i tifosi saranno sempre meno dei cittadini e a un certo punto i cittadini ci lasceranno del tutto.

che declina gli articoli iniziandoli sempre con «*We the People»,* ovvero «Noi, il Popolo», perché le Costituzioni sono non questioncine di palazzo, ma le regole di base che i cittadini si danno. Noi qui dentro, da destra a sinistra dell'Emiciclo, dovremmo ricordarci di essere popolo del popolo e solo in nome del popolo italiano dovremmo agire, far scegliere loro, loro, non temerne la volontà. Così si riporta la gente al voto. Il fine di tutti noi dovrebbe essere chiaro: costruire una democrazia in cui il popolo sia non solo spettatore, ma anche protagonista attivo. La partecipazione vera è nelle urne, non su piattaforme informatiche addomesticate, quella partecipazione della quale qualcuno ha evidentemente paura. Non a caso, da democratici liberali veri, da sempre siamo sostenitori delle preferenze, l'unico metodo di scelta reale del politico da parte dell'elettore, e speriamo davvero che la legge elettorale che accompagnerà questa nostra riforma possa prevederle. Pertanto, mi rivolgo agli italiani per dire loro che ci rende fieri e soddisfatti essere arrivati a questo primo traguardo, che rappresenta una pietra miliare nella storia del nostro Paese: una riforma costituzionale, quella del premierato, pensata soprattutto per dare finalmente stabilità ai Governi di questo Paese, di qualunque colore - sia ben chiaro - per porre Il nostro è l'antidoto più efficace dalla cronica instabilità governativa che ha visto nel nostro Paese alternarsi Governi cosiddetti tecnici, di unità nazionale, di salvezza, patriottici e chi più ne ha più ne metta, lasciandosi dietro solo macerie, lacrime e sangue. Quella messa in campo dal Governo Meloni è una riforma coraggiosa, talmente coraggiosa che non temiamo - anzi la invochiamo - la consultazione popolare, perché ascoltare e confrontarsi con il popolo sovrano è il nostro senso della democrazia. Ci sono voluti più di cinque mesi di incessante lavoro in Commissione e per questo voglio ringraziare il ministro Casellati e il presidente della Commissione affari costituzionali Alberto Balboni, che, con riconosciute competenze e massima disponibilità verso tutti, hanno guidato i lavori permettendo di avere oggi un testo migliore. La verità è che, nonostante una certa opposizione meramente strumentale, tanto in Commissione quanto in Aula, sono state accolte e integrate nel testo proposte costruttive che hanno arricchito questa riforma. Altro che muro di gomma! Altro che Titolo V approvato con tre soli voti di maggioranza! Altro che riforma Renzi in pasto al Paese e sonoramente bocciata, infatti, dal popolo! Totale apertura al dialogo da Governo e maggioranza: questa riforma, infatti, ha attraversato più di 60 sedute di Commissione, con 50 audizioni, 2.600 emendamenti in Commissione e oltre 3.000 in Aula, quasi sessanta ore di discussione generale: numeri che raccontano la verità dei fatti e che fanno riflettere, se pensiamo che i Padri costituenti

si stanno caratterizzando anche in queste ore per essere *contra populi*, volevano abolire il voto, perché secondo loro la democrazia era dannosa, perché i popoli non sapevano votare, ovviamente se non votano a sinistra. se non votano a sinistra. Per noi, viceversa, dare ai cittadini e solo ai cittadini il potere di decidere da chi essere governati, garantendo Governi stabili e affidabili sul piano economico e internazionale, è un impegno assoluto nel rispetto degli italiani. La stagione dei ribaltoni a cui sono state esposte le istituzioni democratiche di questo Paese e a cui purtroppo abbiamo dovuto tristemente assistere nelle ultime legislature possa dirsi arrivata al capolinea. Basta Governi che contraddicono la sovranità popolare espressa nelle urne; basta partiti che perdono nelle urne e poi si ritrovano vincenti al tavolino e al Governo. Già dalla prossima legislatura, infatti, di questo passo potremmo vedere l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Questo significa una sola cosa: permettere quella vera e piena legittimità del *Premier* eletto che in questo Paese spesso è mancata, specialmente con gli ultimi Governi: tra rimpasti *multicolor* e intrighi vari contronatura, la volontà espressa tramite il voto è stata spesso ribaltata, per non dire calpestata. Noi non vogliamo, colleghi, che gli italiani si ritrovino ancora una volta a fare i conti con Esecutivi accozzaglia, privi di indirizzo politico, che si ricordano bene gli italiani che ci ascoltano. Come - statene certi - si ricorderanno bene di chi oggi vuole osteggiare questa riforma con un no preconfezionato e preconcetto, le attuali opposizioni di sinistra, aizzando pericolosamente le piazze, ben consci di infiltrazioni di diverso genere e di manifestare contro la volontà degli italiani in favore di quei poteri dei quali sono maestri. Basti pensare che negli ultimi anni per ben tre volte il PD ha perso le elezioni e per ben tre volte si è ritrovato al Governo. Ecco per cosa manifestate oggi: per la possibilità di governare senza passare per l'investitura popolare. Questo è ciò che volete. Per questo uscite finalmente da quella ZTL e dai salotti al caviale, dove gli italiani vi rimanderanno. Noi, viceversa, crediamo nella squadra italiana, in un'Italia in cui i giocatori in campo sono i cittadini e non le *élite* politiche. Signor Presidente, concittadini italiani, abbiamo dovuto ascoltare ogni menzogna su questa riforma costituzionale, ma oltre ai soliti toni apocalittici, non pare pervenuta alcuna autentica proposta alternativa. Torsione autoritaria, pericolo per la democrazia, sistema plebiscitario, tentativo di forzare un sistema di democrazia parlamentare: sono queste solo alcune delle espressioni che pur autorevoli membri delle opposizioni hanno pronunziato con riguardo a questa riforma, dimenticando pretestuosamente che i principi della riforma altro non sono che i principi connaturali alla stessa storia italiana. L'elezione diretta è radicata nella tradizione politica sin dalla Roma repubblicana e delle città-stato del Rinascimento, imperniata sulla centralità del popolo nella scelta dei propri governanti. Come pure va ricordato che l'Italia è il Paese europeo

perciò rassicurare anche che si è trincerato dietro il Capo dello Stato che, per notizia, è il garante dell'unità nazionale e non un burattino in mano alle sinistre. Non c'è in questa riforma alcuna limitazione delle sue prerogative. Il Capo dello Stato è il nostro organo di garanzia, mantiene tutte le prerogative, anzi gli si aggiunge la revoca dei Ministri. Il Presidente della Repubblica italiana avrà perciò maggiori poteri rispetto agli omologhi Capi di Stato degli altri sistemi parlamentari europei. Questo si tradurrà in maggiore efficienza e responsabilità dell'Esecutivo, naturalmente con dei pesi e dei contrappesi. Mi riferisco in particolare al limite dei due mandati che dovrà avere il *Premier* o la norma cosiddetta antiribaltone, che tanto vi fa orrore. Quanto al potere di scioglimento, certamente ricadrà nelle mani di chi è eletto dal popolo, perché è lui ad avere la fiducia degli elettori, anche se vi dà fastidio; e, quando quella fiducia viene meno, riteniamo giusto ridare la parola al popolo stesso. Questa, signori colleghi, si chiama semplicemente democrazia. Con questa riforma abbiamo anche voluto fortemente riequilibrare la rappresentanza popolare con l'abolizione dei senatori a vita prevista nel testo, proprio per dare il più possibile rappresentanza popolare a tutte le istituzioni. Non ci dimentichiamo infatti che, già prima della riduzione dei parlamentari, la legislatura 2006-2008 si è retta sui senatori a vita; uno scandalo che va in disprezzo della volontà popolare. Chi si distingue per alti meriti si sarebbe dovuto astenere dai voti. *(Applausi)*. Signor Presidente, italiani che ci ascoltate, è del tutto evidente che la parte più importante della riforma costituzionale sia quella che propone di modificare l'articolo 92 della Costituzione, che prevede che l'elezione diretta del *Premier* vincoli il Presidente della Repubblica nell'affidamento dell'incarico al *Premier* votato. Se vogliamo questo, è certamente l'aspetto più innovativo. Già oggi, in verità, quando dalle elezioni emergono un'indicazione chiara del *leader* e una maggioranza di Governo, come è avvenuto in questa legislatura, il Presidente della Repubblica non può che prenderne atto nel rispetto del dettato costituzionale,

degni della stima dei cittadini e della storica grandezza dell'Italia. E lo stiamo facendo, credendo religiosamente che debbano essere i cittadini a decidere chi li governa e non trasformismi di ogni genere. di ogni genere. Lo faremo in sintonia con il popolo sovrano, sapendo che la vostra paura più grande è quella di perdere il treno dei Governi di palazzo. Per dirla come il presidente Mattarella, libertà e democrazia non sono mai garantite. Ecco perché ci battiamo per difenderle sempre e consolidarle, anche con questa riforma.

Signor Presidente, in queste settimane sono stati ampiamente sottolineati i rischi e i limiti di questa riforma, dapprima da parte degli esperti auditi in Commissione e poi anche in quest'Aula, anche dal sottoscritto, dai componenti del mio Gruppo. In questa dichiarazione di voto mi concentrerò dunque, in particolare, sulle conseguenze per le autonomie speciali di Bolzano e di Trento. Negli incontri preliminari con il ministro Alberti Casellati e con il presidente Meloni, ci venne chiesta la nostra opinione sul sistema presidenziale e su quello del premierato. In entrambe le circostanze affermammo che, in linea di principio, non avevamo pregiudizi sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio, purché questa avvenisse in un quadro di contrappesi e bilanciamenti. Eravamo fortemente contrari, invece, al presidenzialismo, perché avrebbe trasformato il Presidente della Repubblica da figura di garanzia a un *totus politicus*, esattamente come in Francia o negli Stati Uniti. Da sempre, ai fini della tutela delle autonomie speciali, la Presidenza della Repubblica è stata una figura fondamentale. Tutte le volte che è montato un sentimento centralista, con richieste e promesse di cancellazione delle autonomie speciali, il Colle ha discretamente fatto presente i precetti costituzionali e gli accordi internazionali che ne sono alla base. È questa la principale ragione, anche se non la sola, che ci spinge a guardare con grande preoccupazione a questa riforma. Un Presidente del Consiglio eletto dai cittadini e un Presidente della Repubblica eletto con i voti della maggioranza di quel Presidente del Consiglio: non più una figura di garanzia, ma un notaio, che vivrà all'ombra del *dominus* del sistema. Signor Presidente, cosa accadrà se torneranno spirare nel Paese sentimenti centralisti, come quelli che, fino a una decina d'anni fa, accomunavano tanti *leader*, forze politiche, anche Presidenti del Consiglio e che tuttora, ogni tanto, affiorano tra le righe di diversi interventi di rappresentanti della politica, anche in quest'Aula? A quale riserva ultima di garanzia potremo appellarci, noi che siamo stati eletti per tutelare e sviluppare le autonomie e per chiedere il rispetto della Costituzione e degli accordi internazionali? Le autonomie saranno costrette a snaturarsi: non più elementi istituzionali e di sistema, non più treno per il Paese destinato a un sempre maggiore decentramento, bensì soggetti in equilibrio precario, tenuti in perenne scacco dal centralismo statale e costretti al corpo a corpo della politica. Non sarà più l'autonomia faticosamente conquistata nei decenni: sarà la sconfitta più grande della nostra autonomia da che esiste. Così come è una sconfitta, ma per l'intero Paese, l'idea che il Senato possa privarsi dei senatori a vita di nomina presidenziale. I senatori a vita sono sempre stati un elemento qualificante del Gruppo per le Autonomie. per le Autonomie, i senatori a vita, da Andreotti in poi, segnalavano il loro profilo istituzionale per tramite di una questione: la tutela delle minoranze linguistiche, che afferisce ai principi base della Costituzione.

Ma non si è voluto farlo, per bassi motivi di convenienza elettorale. Come bene ha detto la nostra Presidente, i senatori a vita sono argomento troppo ghiotto per la probabilmente inevitabile campagna referendaria. L'idea di togliere poltrone all'*élite* piace sempre al popolo elettore, ma, in questo caso, è una contorsione populistica e antipolitica francamente inaccettabile in una rielaborazione della Costituzione. Per restare ancora alle questioni che ci competono come Autonomie, vengo al brutto pasticcio del premio di maggioranza in Costituzione. In questo devo smentire alcuni colleghi dell'opposizione: sono molteplici le Costituzioni che includono riferimenti alla legge elettorale. In Europa, 16 Paesi hanno in Costituzione i principi della legge elettorale e tutti in termini di sistema proporzionale. Ma perché i nostri amici europei sono così affezionati a questo meccanismo, tanto da metterlo in Costituzione? È semplice: semplice: perseguono finalità garantiste, imponendo il metodo elettivo maggiormente equidistributivo e idoneo a rappresentare sempre le minoranze. È l'esatto opposto di quello che viene fatto qui, cioè un premio che prima costruisce e poi blinda la maggioranza, a discapito della minoranza che diventa del tutto impotente. Prendiamo atto e ringraziamo dell'emendamento approvato in Commissione, con cui si ribadisce il principio della rappresentanza delle minoranze linguistiche, che naturalmente, però, dovrà trovare applicazione concreta nella legge elettorale. Ricordo a me stesso che la rappresentanza delle minoranze linguistiche non passa semplicemente dal numero dei seggi per l'Alto Adige, per esempio, ma da una loro attribuzione che rispecchia la proporzione tra cittadini di lingua italiana e cittadini di lingua tedesca e ladina che vivono nella nostra Provincia. Come si andrà a contemperare tutto questo - numero dei seggi, rappresentanza etnica - con il meccanismo del premio di maggioranza, soprattutto in Senato, dove i numeri sono più piccoli? Lo stabilirà la legge elettorale, che avrebbe dovuto, a mio avviso, essere ricompresa in questa discussione sul cambiamento della Costituzione, perché evidentemente sarebbe meglio modificare la Costituzione in funzione della legge elettorale che si intende far approvare al Parlamento, anziché, come si fa qui, riformulare il sistema elettorale in due passaggi slegati tra loro (ora la modifica della Costituzione e domani la legge). Per chiudere, signor Presidente, al netto delle valutazioni più generali già espresse in quest'Aula e soffermandoci su quelle che attengono alle autonomie speciali, è una riforma densa di nubi nerissime. Lo è per i senatori a vita, lo è per la rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche, lo è soprattutto per lo snaturamento delle funzioni e delle prerogative del Presidente della Repubblica; lo è per il futuro, se non per l'esistenza stessa della nostra autonomia. Per questo ci auguriamo che alla Camera, al contrario di quello che è accaduto qui, sia possibile riaprire una discussione vera, accogliendo in consistente parte le buone proposte delle opposizioni, perché mi sento di aver visto un film diverso rispetto a chi mi ha preceduto in questo dibattito. Come lei sa, Presidente, il Gruppo Per le Autonomie comprende senatori di partiti diversi, quindi ciascuno voterà secondo la propria coscienza. Mi sento però di esprimere la convinzione che l'autonomia si tutela portandone avanti con fermezza e serietà i valori e i contenuti e non con i giochi di potere. *(Applausi)*. il Gruppo parlamentare Italia Viva ha chiarito, già in sede di discussione generale, che per noi discutere di elezione diretta del Capo del Governo non era né un'eresia, né un atto di sovvertimento democratico. Abbiamo portato in quest'Aula le riflessioni riformiste di pensatori come Maurice Duverger, Mario Segni, Cesare Salvi, tra gli altri, e le conclusioni della Commissione bicamerale presieduta da Massimo D'Alema, che, nel 1997-1998, immaginò l'introduzione in Italia del premierato. Ci siamo approcciati a questa discussione avendo ancora nelle orecchie e nella memoria, qualcuno penso anche nel cuore, le parole che ci rivolse il 22 aprile 2013 Giorgio Napolitano, al momento della sua rielezione, che cito testualmente: «a esigenze fondate e domande pressanti di riforma delle istituzioni e di rinnovamento della politica

sempre testualmente - che «Non si può più, in nessun campo, sottrarsi al dovere della proposta, alla ricerca della soluzione praticabile, alla decisione netta e tempestiva per le riforme di cui hanno bisogno improrogabile per sopravvivere e progredire la democrazia e la società italiana». È con questo spirito che noi siamo entrati in questo dibattito: scevri da pregiudizi, in maniera laica, con la volontà di contribuire con il nostro pensiero e apportare una visione. Abbiamo presentato, a differenza di altre forze dell'opposizione, un nostro disegno di legge organico, abbiamo avanzato proposte e formulato emendamenti, ma va detto senza infingimenti che il risultato finale è un prodotto deludente, perché, al netto anche di alcuni atteggiamenti (penso a quello della Ministra che in alcune parti hanno fatto rimpiangere un Chinaglia d'annata nei confronti del suo allenatore Valcareggi nel 1974), i nodi sono ancora tutti sul tavolo: il nodo del bicameralismo perfetto, che non avete sciolto; il nodo del ruolo fra Stato e Regioni, che non avete sciolto; il nodo della legge elettorale, che non avete sciolto; il nodo del *Premier* imprigionato dalla ragnatela del diritto di fronda, che avete creato. Insomma, il testo è confuso, disorganico, frutto di compromessi al ribasso tutti interni alla maggioranza e figlio di un clima distante anni luce dallo spirito costituente che dovrebbe informare la riforma della nostra Carta fondamentale. per dirla con una battuta, siamo entrati qui dentro volendo il cittadino arbitro - come ci insegnava Roberto Ruffilli - e rischiamo, con questo testo, di ritrovarci con un cittadino suddito. Per questi motivi, noi non vogliamo concorrere al voto di un errore di questa natura. Si dice che la riforma è una risposta alla crisi della politica. Accettiamo la riflessione, ma entriamo nel merito cerchiamo di comprendere. Scoppola ci diceva che la nostra è una Repubblica dei partiti, che è la specificità di un sistema che era giocato sui partiti e attorno ai partiti snodava il funzionamento della nostra democrazia. Abbiamo attraversato diverse fasi storiche: dalla Prima Repubblica, rigida nella società e bloccata nella democrazia, alla Seconda Repubblica, che - come ha detto Bauman - era una società e una democrazia liquida, vacillante, incerta e fluida, fino ad arrivare a quella che è stata definita la Terza Repubblica, con l'avvento del MoVimento 5 Stelle, funzione gassosa, volatile, cangiante e aeriforme, che ha portato all'oggi, all'evaporazione delle forme della politica, che lascia spazio al vuoto. Non è un caso che, dentro questo mare di cultura politica che si ritrae, emergano antichi ancoraggi da destra e da sinistra. sinistra. La domanda a cui dovremmo quindi rispondere è se siamo davvero davanti al rischio della fine della natura identitaria, strutturale e ontologica della nostra democrazia fondata sui partiti: e, se la fine della democrazia dei partiti è arrivata, da cosa dev'essere sostituita? Da una politica in campagna elettorale permanente? Da *leader* che si fanno *influencer*? Da una ipercomunicazione che viene fatta per colmare l'assenza del pensiero? È per questo, cari colleghi, che noi abbiamo detto che è centrale la legge elettorale. Dobbiamo dire come intendiamo governare il vuoto e declinare la natura identitaria della nostra democrazia; e questa è una risposta che deve arrivare da un processo politico. Ecco l'errore che state compiendo: pensare di risolvere la crisi scaricando tutto sul dato funzionale (la riforma della Costituzione) ed istituzionale (l'elezione diretta del *Premier*). In realtà, i processi politici non possono essere surrogati da geometrie istituzionali e le regole non si possono sostituire alla sostanza del gioco politico. Il punto oggi è capire quali sono le forme della nostra politica, cosa vuol dire partecipazione popolare, quali sono i canali del coinvolgimento democratico, cosa significa far parte di un'associazione per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Cari colleghi, anche alla luce di quello che è accaduto domenica per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, quando 53 italiani su 100 non si sono recati alle urne, non sentite anche voi il senso di vertigine che dà il vuoto che si crea tra il popolo e i suoi rappresentanti, laddove in mezzo non c'è più nulla? *(Applausi)*. Questo è il punto, che si risolve non con un ripristino revanscista e nostalgico di una pretesa età dell'oro che non tornerà più, ma neanche con un appalto fideistico a *leadership* personali. il punto chiave è la ricomposizione fra popolo e Stato ed è questa la cosa che a noi preoccupa maggiormente; è questo il tema al quale ci vogliamo applicare con passione e determinazione, perché - lo sapete anche voi questo testo non è la madre di tutte le riforme. Questo è un rattoppo illusorio, che pretende di chiudere ideologicamente una transizione repubblicana. In realtà, la sfida ineludibile di un'elaborazione strategica e di un'adeguata architettura statuale esige altro dalla subcultura del presentismo, dalle battute via *social* e dalle riletture storiche. È una sfida che quindi esige altro rispetto a questo testo e molto probabilmente, signori del Governo e della maggioranza, esige altro anche rispetto a voi.

Questa che proponete è una riforma dannosa e pericolosa per il nostro Paese, che vuole concentrare il potere nelle mani di una sola persona, riduce le prerogative del Presidente della Repubblica e, assieme all'autonomia differenziata, stravolge la Costituzione italiana. Noi non ve lo permetteremo. Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti che le regole consentono, compreso l'ostruzionismo, che rivendico. Se questo non è stato sufficiente per fermarvi, sposteremo la nostra lotta nel Paese reale. Già oggi pomeriggio qui a Roma, anche per denunciare il clima insopportabile che state montando, e poi in ogni piazza d'Italia difenderemo la Costituzione della Repubblica *(Applausi)*, quella Carta nata dalla Resistenza, nella quale evidentemente non vi riconoscete a sufficienza. La difenderemo nel Paese vincendo il *referendum* confermativo, quando il popolo italiano, come altre volte in passato, si dimostrerà più saggio di chi lo sta governando. Eppure avreste dovuto guardare con più attenzione i risultati delle recenti elezioni europee. Potete nascondervi dietro le percentuali alterate dall'astensionismo, ma poi ci sono i numeri veri, le persone in carne ed ossa. Se avete perso più di un milione di voti in meno di due anni, vuol dire che in tanti stanno comprendendo che il Paese non si governa in questo modo, spaccandolo, lacerandolo e scardinando un punto decisivo su cui sono fondate le democrazie, cioè l'equilibrio dei poteri. *(Applausi)*. Con questa riforma scegliete di marginalizzare definitivamente il Parlamento, ed è proprio questo il vero punto in comune con l'autonomia differenziata. Abbiamo denunciato molte volte lo scambio fatto sulla pelle dei cittadini. Sono due provvedimenti ispirati da logiche che sembrano opposte e che invece insieme prefigurano un pericolosissimo esito: l'autonomia differenziata aumenterà le diseguaglianze; il premierato ridurrà la democrazia e il pluralismo a una contesa plebiscitaria nella quale solo apparentemente i cittadini hanno diritto di scelta. Ci sarebbe stato un modo assai diverso per restituire almeno una parte di quel potere di scelta e si sarebbe potuto fare facilmente, cioè cambiando la legge elettorale e facendone una buona. Avreste dovuto fare questo piuttosto che presentare una proposta in cui il capo del Governo accentra nelle sue mani un potere del tutto squilibrato, senza nemmeno i contrappesi e i bilanciamenti che esistono nei Paesi dove c'è il presidenzialismo. Voi scegliete invece un modello che non ha eguali al mondo e che rischia - caso unico in tutte le democrazie contemporanee - di eleggere il capo del Governo anche senza la maggioranza dei voti con un Parlamento a sua volta eletto, anzi nominato, per trascinamento e ancora più debole di quello di oggi, strutturalmente inadeguato a bilanciare, come invece dovrebbe essere, il potere del capo. Ci dite che c'è un problema di stabilità, che in Italia ci sono stati negli anni troppi Governi: è una questione reale, certamente, che si sarebbe potuta risolvere però senza stravolgere la Costituzione, approvando, per esempio, uno degli emendamenti dell'opposizione sulla sfiducia costruttiva. Non dite una parola invece sull'altra grande questione aperta della nostra democrazia, che ne certifica oggi la crisi profonda, cioè la rappresentanza. Non ne parlate perché evidentemente proprio non la vedete. Ma cosa deve ancora accadere per aprirvi gli occhi? Non basta quello che sta accadendo? Mezzo Paese non va più a votare l'astensionismo cresce dov'è più forte la sofferenza sociale e non si danno risposte ai bisogni reali. È una crisi verticale, che riporta indietro di centinaia di anni le lancette della storia, quando la partecipazione alla vita pubblica non era consentita a tutte le classi sociali. Cosa vogliamo? Una politica che escluda di fatto i poveri, i disoccupati o i precari? Andate a leggere i dati sui quartieri delle nostre città dov'è più alto l'astensionismo e scoprirete che sono loro quelli che a votare non ci vanno più. *(Applausi)*. Dinanzi a questa crisi crisi e al rischio di una così profonda lacerazione sociale, quella che proponete è soltanto una scorciatoia profondamente sbagliata, un rimedio peggiore del male e una torsione plebiscitaria che rischia di fare danni serissimi.

e la progressiva perdita di ruolo del Parlamento, l'abuso dei decreti-legge, il continuo ricorso al voto di fiducia? Ecco, io penso di sì. Il nesso è stato proprio l'inevitabile conseguenza di una tesi sbagliata in radice, cioè il primato della governabilità nei confronti della rappresentanza: con questo avreste dovuto fare i conti. Voi pensate a soluzioni demagogiche. Noi vogliamo ricostruire la democrazia e i pensieri lunghi. Quello che serve è alimentare i canali della partecipazione popolare, ripensare le funzioni della rappresentanza nella direzione di una nuova centralità parlamentare. Serve, in una parola, attuare la nostra Costituzione e non certo demolirla.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, Calamandrei, fautore inascoltato della Repubblica presidenziale, ai tempi dell'Assemblea Costituente previde l'instabilità dei Governi che ha caratterizzato per decenni la Repubblica italiana e auspicò soluzioni più stabili, anche accennando al rapporto tra il Capo del Governo e il Presidente della Repubblica. Dal resoconto della seduta del 5 settembre 1946 della sottocommissione della Costituente, leggiamo disse: «a chi dice che la Repubblica presidenziale presenta il pericolo delle dittature, ricordo che in Italia come si è veduta sorgere una dittatura non già da un regime a tipo presidenziale, ma da un regime a tipo parlamentare (…) in cui si era verificato il fenomeno della pluralità dei partiti e della impossibilità di avere un Governo appoggiato da una maggioranza solida che gli permettesse di governare». «Qual è», si interrogava Calamandrei, «la forma dello Stato che meglio serve a far funzionare un Governo di coalizione, impedendo quelle crisi a ripetizione» - quale capacità profetica, Calamandrei! «che sono la rovina della democrazia (…)?». «Le dittature sorgono non dai governi che governano e che durano, ma dalla impossibilità di governare dei governi democratici» Poi aggiunse: «l'essenziale è che non il Capo dello Stato, ma il Capo del Governo abbia la sicurezza di poter governare». Anche nel 1997, con la bicamerale di D'Alema si ipotizzava un'elezione del Primo Ministro, demandando poi alla legge elettorale i dettagli, al fine di collegarlo a un'ampia base democratica di liste (Cesare Salvi - qualcuno se l'è scordato - fu tra i suoi sostenitori). Qualcuno si è dimenticato anche di questo, pur di sostenere tesi allarmistiche e non basate sulla verità. Siamo al ventesimo mese di legislatura. Tutto si può dire, tranne che questa riforma arrivi in maniera affrettata e prestando il Parlamento. Il Governo, attraverso il ministro Alberti Casellati, che ringrazio per il suo impegno e la sua pazienza, ha avviato molto tempo fa confronti con tutti i Gruppi parlamentari, che hanno portato a modifiche della proposta iniziale. Noi volevamo un presidenzialismo simile al modello americano, poi abbiamo ritenuto che il premierato fosse un punto di approdo che potesse godere di una condivisione più ampia tra le forze politiche. Siamo andati incontro alle proposte altrui senza imporre un disegno predeterminato. Non abbiamo agito con fretta e, pur sapendo che ci attendono numerosi passaggi parlamentari e un possibile *referendum,* abbiamo portato avanti questo confronto. Forse abbiamo atteso anche troppo, perché abbiamo preso impegni con gli elettori. L'altro giorno, in un'intervista a un quotidiano, il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha detto che noi non siamo mai stati chiusi al dialogo, ma l'impegno a fare le riforme lo abbiamo preso con i nostri elettori, non con la sinistra. Allora abbiamo promesso che avremmo lavorato per la riforma della giustizia, della forma di Governo e dell'autonomia, perché vogliamo un Paese più stabile, dove chi investe, chi forma una famiglia o chi pensa al proprio futuro abbia certezze. Il premierato, la riforma della giustizia e la riforma delle autonomie, alla quale tutti abbiamo contribuito, fanno sì che tutte queste riforme aiutino l'Italia. Pensiamo quello che anche Tajani ha ribadito con chiarezza: vogliamo rispettare l'impegno con i nostri elettori. Può sembrare strano a qualcuno, ma noi intendiamo fare La scelta è tra la stabilità o la manovra di palazzo, per un Governo che abbia una base democratica e popolare attraverso le elezioni, come avviene per i sindaci e per i Presidenti di Regione. La scelta, quindi, è tra questa democrazia affidata ai cittadini o l'intrigo (quello che è servito a qualcuno per arrivare al Governo). Abbiamo dato luogo a un confronto ampio, che certamente proseguirà, ma non possiamo subire il diritto di veto. Le minoranze hanno chiesto semplicemente il ritiro della nostra proposta ed è una richiesta antidemocratica, perché si vorrebbe impedire alla maggioranza, frutto di un ampio consenso che si è dimostrato prevalente anche alle elezioni europee, di assumere le proprie decisioni. Non ci arrenderemo al diritto di veto delle minoranze. *(Applausi)*. Per quanto riguarda un tema controverso, i poteri del Quirinale, al Presidente della Repubblica: la Presidenza del Consiglio superiore della magistratura, la nomina dei giudici costituzionali, il rinvio delle leggi alle Camere, l'emanazione di decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti governativi, l'autorizzazione della presentazione dei disegni di legge governativi, la Presidenza del Consiglio supremo di difesa, la ratifica dei trattati internazionali e l'elenco potrebbe continuare, quindi non c'è nessun depotenziamento della figura e delle funzioni del Capo dello Stato. Devo dire che in nessun ordinamento in cui il Presidente della Repubblica non è eletto direttamente dai cittadini, il Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento ha poteri così ampi come quelli che permangono anche dopo l'approvazione del presente disegno di legge. *(Applausi)*. Questa è la verità delle norme, dopodiché la riforma incide sulla prassi al limite dell'ortodossia costituzionale di nominare Governi tecnici o del Presidente a cui, a volte anche per l'instabilità, i poteri dei Presidenti della Repubblica si sono spinti in situazioni complesse. Anzi, il Presidente della Repubblica avrà il potere, su proposta del Presidente del Consiglio, di revocare i Ministri, potere che oggi non ha.

inoltre i colleghi a non essere così rassegnati: quando parlate, date per scontato che noi vinceremo per sempre le elezioni ed eleggeremo il *Premier.* Potrebbe capitare che vinciate anche voi qualche volta,

vogliamo che abbia più spazio la democrazia e non l'intrigo. Nelle ultime ore abbiamo letto con grande allarme l'intervista a una personalità eccelsa di questo Paese, il cardinale Ruini, che ha ricordato come, all'epoca del primo Governo Berlusconi nel 1994, l'allora Presidente della Repubblica invitò perfino i vertici della Chiesa italiana ad agire perché cadesse un Governo nato dalla libera volontà degli elettori. In questo Paese i nemici della democrazia non siedono in questi banchi, ma hanno agito altrove, spesso nell'ombra o a volte con temeraria e pubblica sfrontatezza. Questa è la verità che ha raccontato anche il cardinale Ruini, cari amici.

al ritorno al fascismo, ricordo alcune sortite delle opposizioni anche nelle Aule del Parlamento, alle quali - cari colleghi, qui mi rivolgo più a noi stessi che agli altri - dobbiamo rispondere con il sorriso e con la forza della verità, senza mai cadere in trabocchetti, perché non ci sono situazioni di tensione nel Paese e non ci devono essere nemmeno in queste Aule, quindi dobbiamo rispondere con la forza dei nostri argomenti, che sono a sostegno della democrazia e della libertà del nostro Paese.

genocidi e deportazioni, causando nel XX secolo perdite di vite umane e di libertà di una portata inaudita. Quella risoluzione ricorda l'orrore dell'Olocausto, condanna tutte le ideologie totalitarie come il nazismo e lo stalinismo all'interno dell'Europa e poi chiede una cultura condivisa che respinga i crimini dei regimi fascisti, stalinisti e di tutti gli altri regimi totalitari del passato. Quella risoluzione, signor Presidente, come lei ricorderà, fu approvata convintamente da tanti membri del Parlamento europeo, a partire da quelli del Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia fa orgogliosamente parte, la prima forza politica europea anche oggi dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno.

Questa riforma è per noi fondamentale, perché rafforza la democrazia e la libertà contro ogni tentazione totalitaria ed estremista. Il berlusconismo di cui siamo eredi, ma anche araldi per il futuro, è democrazia diretta, presidenzialismo, riforma della giustizia e valorizzazione dei territori, non facendo scambi, ma riforme per una democrazia più salda e più aperta ai cittadini: più popolo, meno palazzo, questa è la via che indichiamo e per questo votiamo con gioia e convinzione questa riforma. Questa è la verità: più popolo, meno palazzo.

Signor Presidente, Governo, colleghi, inizio dalla fine. Noi voteremo convintamente contro questa riforma, perché siamo convinti che sia sbagliata.

una riforma così importante - abbiamo avuto momenti di acceso scontro in quest'Aula ed è normale che sia così. Le opposizioni si oppongono e la maggioranza giustamente vuole approvare le norme che ritiene opportune per il Paese. Quello che non è stato accettabile è ciò che è accaduto nell'altro ramo del Parlamento, con quel momento di violenza, e ritengo anche inaccettabile che si cerchi di confondere chi è stato aggredito con chi invece ha aggredito,

di dualismo nella maggioranza: c'è chi il Tricolore, come i patrioti di Fratelli d'Italia, lo porta sempre nel cuore e chi evidentemente lo vede come Dracula vede l'aglio. *(Applausi)*. I presupposti di questa riforma, signor I presupposti di questa riforma, signor Presidente, sono assolutamente condivisibili: la stabilità, il rispetto della volontà popolare e il tentativo di frenare i ribaltoni.

possono non stimolare il passaggio da un Gruppo all'altro. Guardate infatti che governabilità, stabilità, rispetto della volontà popolare e blocco dei ribaltoni non si fanno per legge,

laddove avesse i quattro voti delle Assemblee del Parlamento e l'approvazione referendaria, non garantirà in nessun modo che il secondo *Premier* eletto nelle file di una maggioranza non possa cambiare la maggioranza parlamentare dopo aver avuto il reincarico. Non c'è scritto da nessuna parte che questo sarà vietato. L'unica cosa che c'è scritta è che casomai, se due Presidenti del Consiglio saltano, per un motivo o per l'altro, si torna al voto, anche se non c'è un motivo politico per cui i Presidenti debbano lasciare il proprio incarico. Anche questo è un assurdo: il fatto che ci sia la previsione di uno scioglimento delle Camere senza una motivazione politica è un assurdo costituzionale, che voi costituzionalizzate. La dinamica di elezione del secondo *Premier* è, quella sì, la costituzionalizzazione del ribaltone, perché in qualche modo si daranno le chiavi del Paese a qualcuno che, anche in una Costituzione che prevede l'elezione diretta, non è stato eletto direttamente. Quello non è un ribaltone?

State sfruttando questo momento di consenso - che è lecito ed esiste, perché sono onde che accadono - per modificare gli assetti complessivi dello Stato

per evitare che poi ci sia un percorso democratico che possa riaccendere un dibattito veramente democratico nel Paese. Questo è ciò che state cercando di fare. Autonomia differenziata, da un lato, premierato, dall'altro, e riforma della giustizia costituiscono un disegno molto chiaro: volete concentrare il potere nelle mani di un'unica persona, sulla base di un'investitura popolare che dovrà poi confrontarsi con un Presidente della Repubblica che quell'investitura non ce l'ha. A scanso di equivoci, vorrei dire a chi dice che non vengono toccati

Voi concentrate sul Presidente del Consiglio eletto ogni tipo di potere. Ricordo la riforma della giustizia fatta contro la magistratura la separazione delle carriere; il passaggio successivo sarà evidentemente un ridisegno dell'obbligatorietà dell'azione penale, cui il Parlamento dovrà decidere (questa è la grande visione della giustizia, in particolare di una forza politica della maggioranza). Ricordo poi l'autonomia differenziata, che spacca il Paese e non fa il male del Sud e il bene del Nord, ma il male delle aree interne e più povere, dove c'è maggior degrado, che siano al Sud, al Nord o al Centro.

Tornate a una proposta sul presidenzialismo e facciamo una discussione seria in merito. Noi siamo contrari, ma almeno ha un senso per il rispetto del vostro elettorato, che vi ha votato per un programma elettorale che prevedeva l'elezione diretta del Presidente del Repubblica. Ha un senso perché è un modello che funziona in altri Paesi. Ripeto che non è il nostro modello, né il mio, né della mia forza politica, ma ha un senso costituzionale più alto della riforma che state facendo oggi. che state facendo oggi. È evidente che siamo in un contesto in cui, se facciamo l'opposizione, è perché non abbiamo i numeri in Parlamento per bloccare qui in queste Aule la riforma Fuori da queste Aule però, a partire da oggi, dove ci confronteremo con la piazza, c'è un Paese che vuole esprimersi su questo tema. Lo farà nella dinamica referendaria e sono convinto che lo farà consapevolmente, bocciando questa riforma: sarà l'inizio del vostro declino politico. *(Applausi)*. Signor Presidente, iniziamo la nostra dichiarazione di voto sottolineando che una delle critiche più forti durante la discussione generale su questo argomento, la riforma costituzionale inerente all'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, è arrivata dalle opposizioni, con riferimento allo scambio

Qui si parla di accordo politico tra forze di maggioranza, che hanno tutto il diritto di farlo *(Applausi)* e, anzi, tengono unita questa maggioranza e l'hanno tenuta unita anche in passato. Non dimentichiamo, infatti, che queste riforme

L'attinenza e le similitudini, però, sono assolutamente totali. In quella riforma c'era comunque un primo passo verso il federalismo e una sua piena attuazione: c'erano la famosa devoluzione dei poteri dallo Stato alle Regioni sui temi della sanità, dell'istruzione e della polizia locale; l'istituzione del Senato federale, che coinvolgeva direttamente i territori; la ridefinizione dei poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica; la modifica della composizione della Corte costituzionale e anche del Consiglio superiore della magistratura, proprio per superare il cosiddetto tema delle correnti di giustizia. Anche in quell'occasione quindi, nel 2005, in quella riforma voluta da tutto il centrodestra, con la Casa delle Libertà, era di fatto previsto il sostanziale rafforzamento del potere esecutivo e, più specificamente, del Presidente del Consiglio dei ministri,

pura e semplice, disciplinata dall'articolo 94 della Costituzione, conduceva alle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri e allo scioglimento automatico delle Camere. Tutto molto simile quindi, come vi ho detto, a quello che oggi il centrodestra ripropone, naturalmente con tre riforme differenti. È la coerenza del centrodestra che ci fa perseverare nell'obiettivo di raggiungere determinate riforme.

posso dirlo meglio: diciamo che per il centrosinistra l'autonomia è buona se il centrosinistra governa, ma diventa cattiva se il centrosinistra va all'opposizione. Non ci dimentichiamo le proposte di maggiore autonomia, con tante richieste di materie, così come previste dalla Costituzione, fatte dal presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini *(Applausi)*, dall'allora vice presidente della Regione Emilia-Romagna, attuale segretario del Partito Democratico, Elly Schlein *(Applausi)*, dal presidente De Luca, che nel primo Governo giallo-verde correva dalla già ministra Stefani per chiedere più autonomia dei territori. Me lo ricorda sempre il collega Cantalamessa: ci sono tante dichiarazioni ben scritte e ben chiare, come a dire che ai tempi anche la Campania riteneva che l'autonomia fosse assolutamente utile al territorio, perché alla fine è proprio così. Altro che scardinamento dell'architettura costituzionale. Con l'autonomia valorizziamo i territori nel nome di un principio dell'unità delle diversità, che sarà il vero collante di un Paese oggi profondamente diviso. Con il premierato diamo stabilità al Governo per evitare quei ribaltoni che i cittadini non hanno mai tollerato. Insomma, ai maggiori poteri che diamo al Presidente del Consiglio dei ministri, come bilanciamento, daremo più poteri ai territori. Era il giusto bilanciamento a tutela e a garanzia dell'unità del Paese.

la palla passerà fondamentalmente alla Camera -, se penso ad alcune obiezioni, per esempio sollevate dal presidente Pera, circa i contrappesi da aumentare e allo statuto dell'opposizione da introdurre, molto dipenderà - noi lo diciamo - dall'eventuale disponibilità del Gruppo di Fratelli d'Italia, che ovviamente spinge molto su questa riforma, di apportare miglioramenti e accorgimenti, togliendo magari qualche freccia dall'arco delle opposizioni in vista del *referendum* confermativo, visto che, insomma, i precedenti non hanno sicuramente portato molto bene. Ma dipenderà anche molto dalle stesse opposizioni,

naturalmente il testo, a prescindere da quella che può essere una valutazione complessiva della riforma, che sappiamo sarà comunque a vostro giudizio negativa. Quello che invece è certo è che da parte della Lega ci sarà il massimo rispetto di questo accordo politico, perché la credibilità di un partito politico e di un politico in generale si misura dalla sua capacità di rispettare i patti, gli accordi e la parola data *(Applausi)*, motivo per cui esprimiamo a nome del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'azione il voto favorevole a questa riforma costituzionale.

prerogative democratiche, a batterci per farvi cambiare idea, ma dopo aver sentito i Presidenti dei Gruppi di maggioranza, per il momento Gasparri e Romeo, è evidente che, nonostante i lunghi silenzi dei Gruppi di maggioranza, non siamo riusciti a far cambiare idea sugli aspetti principali che sottoponiamo oggi all'attenzione dell'Assemblea e, attraverso la diretta televisiva, anche a chi ci ascolta da casa. Presidente, la Costituzione non ha e non può avere né un'ideologia, né una filosofia di parte»: queste sono le parole di una Madre costituente, signora ministra Casellati, una madre autorevole, Nilde Iotti, che non a caso, da Costituente, ricordava a tutte e a tutti in quel tempo che la Costituzione non era di parte e se c'era una certezza nella nostra Carta costituzionale, allora come oggi, era quella connessa alla cultura della convivenza con lo sforzo di riconoscere le identità di tutti senza arrendersi di fronte alle diversità. Voglio dirlo con chiarezza ai colleghi e alle colleghe della maggioranza: identità di tutti, senza arrendersi di fronte alle diversità. Abbiamo fatto ogni sforzo per non arrenderci all'evidenza di quello che è apparso, sin dal primo momento, un indegno baratto politico. Altro che scambio, presidente Romeo; questo è stato un baratto politico. La democrazia, così come è stata concepita nella nostra Costituzione, è il tentativo di avere porte aperte. Porte e possibilità aperte a cosa? Alle trasformazioni sociali, a trasformazioni che accompagnano l'evoluzione della società, non che la frenano. E mi riferisco soprattutto alla veemenza con cui rappresentate - ed è la cosa che più ci preoccupa di questa proposta di riforma - i principi di identità e di nazionalismo alla base della proposta politica della destra, che, in nome di una presunta efficienza decisionale (che è emersa ancora oggi), chiede più poteri nelle mani del Presidente del Consiglio. Ma non vi sono bastati, in venti mesi, 65 decreti-legge e quasi 50 voti di fiducia messi contro voi stessi? Non vi basta questo potere, ne volete di più? Non avete mai ricercato il consenso comune, in questi venti mesi; consenso che deve essere sempre e solo ritenuto prossimo al bene sociale, non al bene di una forza politica. Presidente Romeo, presidente Gasparri, presidente Malan, voi pensate al bene della singola forza politica e giustificate quello che noi chiamiamo baratto come un accordo elettorale. Quella roba lì è fatta sulla pelle del Paese, sulla pelle della Costituzione. Come hanno sottolineato in Commissione in tutti questi mesi i colleghi Parrini, Giorgis (il nostro Capogruppo, che ringrazio), Valente, Meloni e tutto il Gruppo Partito Democratico, avete deciso di limitare e ridurre la democrazia partecipativa e pluralista, fondata sulla separazione dei poteri, all'elezione diretta del *Premier*, con l'elezione di una sua maggioranza parlamentare eletta per trascinamento; esattamente l'opposto di quello che in quest'Aula poco fa ha detto il presidente Gasparri. L'Italia passa, con la vostra proposta, dalla primazia del Parlamento alla primazia del Governo. In questa bulimia di potere, signor Presidente, lei ha provato a costruire un campo di gioco rispettoso delle regole, anche se la tagliola - come le abbiamo detto più volte - poteva farla scattare qualche seduta dopo. Ma la maggioranza ha provato a far passare uno scambio politico tra le sue forze garantendo irresponsabilmente ad ognuno un pezzo di vita del Paese. Quello che il presidente Romeo chiama federalismo, si chiama spacca Italia *(Applausi)*; non ci sono i LEP, presidente Romeo, non ci sono i livelli essenziali delle prestazioni, le diseguaglianze restano le stesse sul trasporto pubblico locale, sulla sanità, sulla scuola e sull'assistenza, dai bambini agli anziani. Non se lo dimentichi, presidente Romeo, perché poi risponderete agli italiani. *(Applausi)*. Così come l'asservimento al Governo del potere giudiziario e i pieni poteri alla presidente Meloni.

non merita le offese del presidente Gasparri. *(Applausi)*. Allo scambio politico inaccettabile si aggiunge un atteggiamento aggressivo da parte della destra, come è accaduto qualche giorno fa alla Camera, con una vera aggressione ai danni dell'opposizione, semplicemente per aver esposto un tricolore. La bandiera, colleghi, non è una provocazione - come invece ha detto la presidente Meloni - ma il messaggio di chi difende sempre sempre - e ribadisco sempre - la Costituzione antifascista che si fonda sulla convivenza tra diverse identità. *(Applausi)*. Per questa ragione saremo in piazza Santi Apostoli più tardi, dopo il voto qui in Aula, per dire no, e ancora no (e continueremo a dirlo) al baratto tra autonomia differenziata e premierato. Ma sono passati venti mesi, presidente La Russa. In venti mesi di Governo abbiamo

5 milioni all'inizio degli anni Novanta. È una responsabilità collettiva di tutti i Governi che si sono succeduti. Abbiamo un problema serissimo di calo demografico: una Provincia su tre in Italia ha più pensionati che popolazione attiva. Mentre il mondo passava da 4-4,5 miliardi di popolazione complessiva negli anni Ottanta l'Italia è passata da 60 milioni nel 2015 a 58 milioni oggi. Negli ultimi tredici mesi le imprese hanno registrato una variazione tendenziale negativa.

con un Governo che anziché rispondere ai temi che pongono ogni giorno i sindacati, le imprese, le associazioni di volontariato, le associazioni che ogni volta consentono al nostro Paese di resistere, o nasconde la verità, come ha fatto con il DEF, o mente. Signor Presidente, potremmo continuare: potremmo ricordare le tasse chiamate "pizzo di Stato"; potremmo ricordare i diciannove condoni, compreso l'ultimo varato dal vice presidente Salvini; potremmo ricordare "l'erroraccio" sul redditometro. Questo siete stati in questi venti mesi. *(Applausi)*. Anziché rispondere ai problemi degli italiani, venite qui e il problema che ponete davanti al Paese è la Costituzione repubblicana?

per cambiare la Costituzione, signor Presidente. La cambiate contro la sinistra che si oppone, contro i giudici che indagano, contro gli studenti che manifestano, contro gli intellettuali che obiettano, contro i giornalisti che scrivono. Voi pensate che davvero quello che stiamo dicendo qui lo pensano il PD e i partiti di opposizione? È un giudizio unanime che va dai giuristi ai costituzionalisti, dalle parti sociali alla Chiesa. Siete stati addirittura costretti ad attaccare la CEI e il cardinale Zuppi *(Applausi)*, colpevoli di dire che il re è nudo e che quel papocchio di presunte riforme rischia di minare le basi di quel vincolo di solidarietà che è presidio dell'unità della Repubblica. la ringrazio davvero per quest'ultimo minuto che mi dà a disposizione. Quella cultura unitaria della convivenza trova una naturale forma nella celebrazione della dignità, dell'identità. La vostra politica dell'identità maggioritaria alimenta solo una forma aggressiva di nazionalismo che non ci porterà da nessuna parte. Quello della convivenza di ogni identità - concetto che dovremmo aver presente - è il Il pericolo che sentiamo è che si stia trasformando una sorta di egemonia etnica che cancella la parità dei diritti e mina l'unica identità nazionale condivisa, che è quella antifascista, in una idea di Paese che non ci piace e che combatteremo. Noi e il Paese - ha detto Liliana Segre in un bellissimo intervento in discussione generale sulla riforma costituzionale - non possiamo e non vogliamo tacere, e non lo faremo.

L'Italia ha un problema di stabilità che ci portiamo dietro dalla notte dei tempi e che si traduce con una durata media dei Governi di un anno: 414 giorni per l'esattezza. Tale problema di stabilità, visto che qualcuno che qualcuno lo vuole ignorare, secondo dati del «Sole 24 ore» è costato negli ultimi dieci anni 265 miliardi ai cittadini italiani.

ha un costo e noi ci siamo assunti la responsabilità di risolverlo con una proposta che certo, come qualcuno ha detto (anche il collega Franceschini) forse non ci conviene. Certo, è una proposta rischiosa, ma noi non volteremo mai le spalle ai cittadini italiani per non affrontare il rischio di risolvere un problema dell'Italia. Lo dico chiaramente perché il 9 maggio 2023, la presidente il 9 maggio 2023, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato tutte le opposizioni, partendo da una proposta di di presidenzialismo che era quella che voleva portare avanti il centrodestra per risolvere il problema della stabilità e, incontrando tutte le opposizioni, ha proposto una soluzione di mediazione. Alcune forze di opposizione hanno deciso di partecipare in maniera costruttiva, magari anche non condividendo questa proposta, alcune avanzando una loro proposta di premierato ancora più spinta rispetto a quella che abbiamo presentato. Il 9 settembre ci sono state alcune forze di opposizione che hanno deciso di chiudere la porta a qualsiasi proposta. Ci sono tre forze di opposizione che legittimamente hanno deciso di non partecipare a un percorso di condivisione e di risoluzione del problema della stabilità, seguendo il "l'elezione diretta non s'ha da fare" e del "no al presidenzialismo", "no al premierato", non sono una priorità per il Paese. Il premierato non s'ha da fare. s'ha da fare. Quel giorno, quando queste forze hanno scelto di speculare sulla riforma costituzionale, dico molto chiaramente che non sono state voltate le spalle al Presidente del Consiglio, sono state voltate le spalle agli italiani *(Applausi)* che, in assenza di una riforma, dovrebbero continuare a pagare l'instabilità del Paese. È questo che non è accettabile. Da qui l'ostruzionismo che è stato fatto in Commissione e in Aula, le provocazioni, gli insulti, la ricerca costante di uno scontro che in quest'Aula non è stata raccolta. non è stata raccolta. Da qui anche le continue interruzioni quando noi interveniamo, perché il premierato - va detto chiaramente ai cittadini italiani - altro non è che quello che già accade in altri Paesi, ma soprattutto nei Comuni, dove i cittadini scelgono i sindaci e i sindaci hanno una maggioranza che consente loro di governare; è quello che accade nelle Regioni, dove i cittadini scelgono i governatori e i governatori hanno una maggioranza che consente loro di governare e che dà loro stabilità. È quello che accade anche in altri Paesi come il Regno Unito, che è stato citato e che non mi pare, come ricordava il collega Pera, un pericoloso Stato

PRESIDENTE. Non ho avuto bisogno di intervenire per lasciar parlare tranquillamente nessuno. È la prima occasione oggi in cui c'è un disturbo di fondo. Vi prego di lasciare esprimere la propria opinione al senatore Lisei senza mugugni di fondo, grazie. non potrà più nominare i senatori a vita, avrà qualche grattacapo in meno e non dovrà più intervenire per risolvere i problemi causati dall'instabilità della politica. Senatrice Malpezzi, la vedo agitata oggi. tutto e il contrario di tutto, le vostre affermazioni sono state un'offesa alla coerenza: volete il sistema parlamentare tedesco, però non volete gli Stati federali; vi piacciono le elezioni americane di *midterm*, ma vi piace anche che il

è che non è stata presentata una proposta alternativa. PRESIDENTE. Non capisco il tentativo di impedire di esprimere un'opinione che non è assolutamente diversa da quella di segno opposto che abbiamo sentito in tutto il dibattito. Prego, senatore La verità è che l'unica proposta alternativa è stata quella presentata dal Gruppo Italia Viva e anche da altri Gruppi che hanno inteso partecipare

ha modificato il Titolo V e se ne è pentito, ha fatto le leggi elettorali con le liste bloccate e se ne è pentito, ha promosso e votato la riforma Renzi-Boschi e se ne è pentito. Vi siete pentiti di qualsiasi cosa abbiate fatto, siete il partito dei pentiti costituzionalisti, quindi non accettiamo lezioni di costituzionalismo da voi.

Non accettiamo neanche lezioni di rispetto delle istituzioni, come dimostrano queste interruzioni e i tanti atteggiamenti che ci sono stati nel corso del dibattito,

soprattutto, respingiamo ogni ricostruzione fantasiosa di un possibile pericolo fascista, che è inesistente, anche perché i richiami alla legge Acerbo sono completamente sbagliati,

a non accettare l'ordine dei lavori, ma l'ultimo degli interventi è quello del partito più grande, dovete avere la consapevolezza che non va interrotto solo perché è l'ultimo. Prego senatore Lisei, prosegua, potrà recuperare il tempo perso. Troviamo che siano delle speculazioni in malafede i continui richiami a un pericolo fascista o a una torsione autoritaria, capisca che il caldo tepore del pericolo fascista possa riscaldare il freddo inverno delle idee della sinistra, ma purtroppo questo progetto di legge…*(Commenti).* PRESIDENTE. Senatore Sensi, la richiamo all'ordine. Senatore Lisei, non dica "voi", si rivolga a me quando interviene. Grazie dell'applauso, ma non può essere selettivo solo quando vi fa piacere: o c'è sempre o non c'è mai. Una delle critiche principali che è stata fatta è che questo sistema ce lo avremmo solo noi. Lo capisco, credo che le riforme costituzionali siano come un abito e vadano calzate anche sulle esigenze della Nazione e

dico anche che la nostra è l'unica Nazione nella quale, quando c'è un'emergenza nazionale o quando c'è una crisi internazionale, siamo costretti a stringerci tutti intorno a un banchiere o a un tecnico, perché non ci si può stringere intorno a un Governo politico e credo che questa sia un'altra anomalia. la nostra è forse l'unica Nazione nella quale arriva e diventa Presidente del Consiglio una persona completamente sconosciuta dal resto degli italiani, mai votata e mai eletta. Abbiamo delle anomalie e la volontà è ovviamente di risolverle e di evitare che accadano nuovamente certe cose. Dico molto banalmente, in conclusione, che la cosa che mi fa più arrabbiare è che le argomentazioni che sono state usate nel corso le argomentazioni che sono state usate nel corso del dibattito sono soprattutto e restano un'offesa al popolo italiano. *(Commenti).* sostenere, come è stato fatto, che gli italiani siano abbastanza intelligenti per votare il sindaco, per votare il governatore, per pagare le tasse, per pagare il superbonus, ma non lo siano per scegliere il Presidente del Consiglio

che è quello che ho anche richiamato prima in qualche passaggio, che è Alessandro Manzoni, che diceva - credo giustamente - che si dovrebbe forse pensare più a far bene che a star bene e così forse si finirebbe tutti per star meglio. Con questa riforma l'Italia starà meglio.

Allora è stato dato, come ho annunciato, un minuto in più per le interruzioni; esattamente lo stesso tempo in più che ho dato senza interruzioni all'oratore del Partito Democratico. *(Applausi)*. Controllate gli orari e impariamo, per favore, ad essere almeno

prendo la parola solo per pochi secondi per esprimere il voto in dissenso dal Gruppo in rappresentanza della componente SVP alla quale appartengo. La riforma orientata all'accentramento dei poteri del Governo centrale potrebbe rappresentare delle criticità per noi appartenenti alle minoranze linguistiche. linguistiche. In caso di entrata in vigore della riforma costituzionale che ci accingiamo a votare oggi in prima lettura, come facilmente immaginabile, diventerà assai più importante l'attenzione che il Governo centrale e la relativa maggioranza presteranno ai temi delle minoranze linguistiche e ai loro rappresentanti in Parlamento. Il ministro Casellati e il presidente Balboni hanno compreso la nostra preoccupazione e li ringrazio per aver accolto nell'articolo 5 un principio per noi molto significativo ossia quello che prevede direttamente in Costituzione, accanto al principio di rappresentanza, anche quello di tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del premio di maggioranza. Naturalmente il principio dovrà poi trovare concreta attuazione anche nella prossima legge elettorale; motivo per cui noi, come SVP, allo stato esprimiamo un voto di astensione.

«Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica». Prima di dichiarare aperta la votazione, voglio comunque ringraziare tutti i senatori per avere oggi, sia pure in un momento di appassionato confronto e dibattito, mantenuto complessivamente un clima di civiltà che fa loro onore. Grazie. *(Segue la votazione).*

ha avuto un gravissimo incidente, addirittura con un braccio tranciato durante il suo lavoro. Questo lavoratore, che ha subito anche dei gravi incidenti ha dei problemi alle gambe, anziché essere aiutato dal suo padrone, dalla persona per la quale lavorava...

Questo lavoratore, che ha avuto appunto un incidente gravissimo, anziché essere aiutato ad andare in ospedale, per provare, anche *in extremis*, ad essere curato, è stato scaricato come un vero e proprio rifiuto dal suo padrone di lavoro in condizioni gravissime. Io penso che quanto avvenuto sia di una gravità estrema, che si tratti di un vero e proprio orrore, di vera e propria schiavitù, che ha molto a che fare con un approccio mafioso al caporalato.

dello sfruttamento costante che questi lavoratori subiscono e anche di realtà che sono, dal punto di vista giudiziario, da verificare. Credo di avere letto che c'è già stata l'apertura di un'inchiesta, di un'indagine. Però, io non mi vorrei limitare al lavoro, seppur doveroso, della magistratura, ma piuttosto vorrei avviare una riflessione a tutto tondo su queste forme di sfruttamento e su questa forma di disumanità. Per questa ragione, signor Presidente, le chiedo di convocare una seduta del Senato per discutere di questi temi. Chiederò anche alla Commissione antimafia di esprimersi, perché qui dentro c'è anche un tema che riguarda il fatto il fatto che alcune di queste realtà sono realtà che sfruttano in modo mafioso questi lavoratori. Chiedo di non sottovalutare in alcun modo questo tema, perché io penso che se le nostre coscienze non sono in grado di osservare un secondo di silenzio

Presidente, la invito a prendere in considerazione la nostra richiesta, perché davvero quello che è successo ieri, secondo me, va molto oltre ogni possibilità di accettare qualsiasi tipo di approccio al tema del lavoro.

Signora Presidente, intervengo per chiedere un'informativa in Aula del ministro Nordio per la situazione tragica delle nostre carceri. fine settimana ci sono stati altri quattro suicidi; tra l'altro, uno dei quattro detenuti che si è suicidato aveva settantasette anni ed era ancora detenuto. Abbiamo una situazione terribile: i suicidi dall'inizio dell'anno sono 44, il che fa di quest'anno, se il dato fosse proiettato fino alla fine dell'anno, con la stessa costanza di un morto praticamente ogni tre giorni, il peggiore di questa catena di morti che dobbiamo fermare. Non è un caso, signora Presidente, se ci troviamo davanti a questo stillicidio di vittime. È il frutto di una situazione carceraria insopportabile, intollerabile, non degna di un Paese civile: nelle nostre carceri ci sono 15.000 detenuti, più di quanto esse potrebbero contenere. Aumentano i numeri dicono le statistiche - di 330 nuovi carcerati al giorno. Questo ci esporrà quasi certamente a una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, che già ci vide, con la famosa sentenza Torreggiani, oggetto di una censura internazionale. Allora qui, tenendo conto anche che andiamo verso la stagione estiva, le nostre strutture fatiscenti sovraffollate rendono la permanenza delle persone che sono incarcerate ancora più intollerabile, bisogna trovare una soluzione. Noi chiediamo innanzitutto al Ministro di venire in Aula a spiegarci che cosa sta facendo il Governo e come intende interrompere la catena di morti. Voglio ricordare che in Commissione giustizia alla Camera si sta discutendo una proposta di legge a prima firma dell'onorevole Giachetti sulla liberazione anticipata e noi auspichiamo naturalmente che venga approvata. Chiediamo però che il Governo, innanzitutto, agisca molto rapidamente, perché qui parliamo di un tributo di vite umane che - ripeto - non è più accettabile, e prenda immediatamente delle misure. Deve poi informare il Parlamento di quello che succede nei nostri penitenziari, che sono una parte del Paese e non discariche di rifiuti, dove mettiamo gente di cui non sappiamo cosa fare e che poi non vediamo, mettendoci così a posto la coscienza. Quella è una parte dell'Italia e il Governo deve prendersene la responsabilità. Quindi, le chiedo, per favore, di trasmettere al Governo la richiesta che il ministro Nordio venga quanto prima in Aula a informarci sulle azioni del Governo per interrompere questa situazione, che - ripeto - è intollerabile.

fare anch'io un intervento accorato. Ci siamo già prima in Commissione giustizia, assieme al senatore Scalfarotto, confrontati sul tema e non so se posso usare questo termine: non è una richiesta politico-partitica, ma è una richiesta civile. Quello che sta succedendo non è un problema che riguarda solo una parte di quest'Aula o del Parlamento: è un tema che riguarda tutti, che indigna e preoccupa tutti in maniera drammatica. Che altro deve succedere perché ci sia un sussulto di tutti, maggioranza e opposizione, su questi temi? Io dico sempre - e non cosa che non abbiamo fatto in tutti questi anni, in carceri più umane, in carceri che rispettino l'articolo 27 della Costituzione: pena certa, anche alternativa, ma tesa alla rieducazione e al reinserimento. Ebbene, chi investe su queste cose poi investe in sicurezza, perché un detenuto che, dopo aver scontato la pena, esce rieducato non torna a delinquere. Oggi in Commissione abbiamo anche chiesto e ottenuto qualche disponibilità di massima che venga anche un altro soggetto a dirci cosa fa: il Garante

una è riservata alla Commissione giustizia, ma la voglio esplicitare anche qui ed è stata condivisa; l'altra è avere il Ministro a parlare alla Camera - come è già stato chiesto - e anche qui in Senato, della situazione delle carceri. È davvero un dovere civico, prima ancora che istituzionale e politico.

che manifestava intenti suicidari all'interno di una stazione di servizio, su una strada ad alta intensità veicolare e a scorrimento veloce, quale la 16-*bis*; dall'altra parte, l'atto eroico di due poliziotti, Orazio Pugliese e Francesco

tra i veicoli. Perché questo episodio, che per me ha una pregnanza notevole? La malattia mentale molto spesso è connotata dalla cultura dello scarto, dall'indifferenza,

come dovrebbero e che invece hanno messo a repentaglio la loro vita per salvarne un'altra. Questo per me, che appartengo a una cultura cattolica che porta in evidenza il valore della vita, è stato un gesto molto significativo. penso sia stato utile che in quest'Aula si sia data notizia e che resti traccia di un gesto eroico che segna